La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 dicembre. Questa mattina sarà discusso il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la continuità del servizio scolastico. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi è integrato con 1'esame - a partire dalle ore 16,30 della proposta concernente l'inserimento nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza della XVI legislatura. Si ricorda che per la votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. A conclusione del voto - sempre oggi pomeriggio - potrà riprendere la discussione del decreto-legge sul servizio scolastico, ove non concluso. Il calendario della settimana corrente è inoltre integrato con il disegno di legge sulla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. La prossima settimana - dal 24 al 26 novembre - è previsto l'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia di lavoro pubblico e privato, nonché di ratifiche di accordi internazionali e di mozioni da definire. Per quanto riguarda la definizione degli argomenti oggetto delle mozioni, con particolare riguardo a quelle sollecitate dai Gruppi di opposizione, si è convenuto di riconvocare in settimana la Conferenza dei Capigruppo. Nella seduta pomeridiana di giovedì 26 novembre saranno svolte interrogazioni a risposta immediata sul lavoro notturno del personale femminile della CAI S.p.A. e sull'utilizzo dei fondi per il dissesto idrogeologico con particolare riguardo all'alluvione di Messina. Nella settimana successiva alla prossima - dal 1° al 3 dicembre - sarà discusso il decreto-legge recante proroga di missioni internazionali. Il calendario prevede inoltre 1'esame di disegni di legge fatti propri dalle opposizioni recanti introduzione del reato di tortura nel codice penale, nonché mozioni, anche queste da definire. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il calendario potrà essere integrato con il disegno di legge in materia di contabilità e finanza pubblica, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ove concluso dalla Commissione competente.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 1835, recante conversione in legge del decreto-legge n. 134, già approvato dalla Camera dei deputati, scade il 23 novembre prossimo, quindi è a rischio decadenza. Questo è il motivo della sua sostanziale blindatura (la maggioranza proverà a blindare questo provvedimento) e forse anche il motivo delle diverse strategie con cui approdano in Aula maggioranza e opposizione, che pure hanno condiviso le tante luci del provvedimento, rilevando altresì alcune ombre delle quali cercherò di tenere informata l'Assemblea. Il decreto dispone - nel più generale contesto della riforma organica della scuola, del razionale utilizzo delle risorse e del miglioramento della qualità del servizio la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie previste anche ai sensi della legge finanziaria 2009. quindi il problema di circa 15.000 precari con contratto a tempo determinato, titolari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Esso dispone che, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010, l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta, ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti. Tali assegnazioni preferenziali avvengono anche per quel personale che nell'anno scolastico 2008-2009 abbia conseguito una supplenza per almeno 180 giorni. In tale contesto vanno viste anche le intese con le Regioni con le quali attivare progetti di carattere straordinario anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento, si prevede che, a partire da biennio 2011-2012 e 2012-2013, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie avvenga sulla base del principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento in altra Provincia con l'inserimento in graduatoria con il punteggio precedentemente maturato. Voglio inoltre far riferimento alla norma introdotta dalla Camera dei deputati relativa all'applicazione della legge n. 104 del 1992. La disciplina introdotta non intende in alcun modo vessare categorie svantaggiate ma, al contrario, tutelarle da eventuali abusi. Vi è poi la

dell'articolo 1. Questo comma, che è stato inserito nel provvedimento dalla Camera dei deputati,

il Presidente della Repubblica non vede di buon occhio l'approvazione di questo comma. Quindi, possiamo dire che la maggior parte delle obiezioni dell'opposizione - peraltro, ripeto, nel merito condivise - si fermano a tale aspetto. C'è poi una posizione dei colleghi della Lega che manifestano perplessità in merito all'inserimento a pettine nella graduatoria per quanto riguarda l'aggiornamento delle graduatorie nel biennio 2010-2011 e 2011-2012. Credo però, signor Presidente e colleghi, che mentre noi affrontiamo - e bene - il problema di circa 15.000 precari, dimentichiamo che la pletora dei precari è di circa 570.000 unità: sono infatti 270.000 i precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e 300.000 i precari senza abilitazione inseriti nelle graduatorie di istituto. Credo che il Governo abbia il dovere di dire una parola chiara a questi docenti precari,

quindi il dovere di dire a costoro una parola di chiarezza su che cosa vogliamo fare e quando pensiamo di affrontare e risolvere i loro problemi. ho ritirato gli emendamenti a mia firma, contenuti nel relativo fascicolo, e ho presentato un apposito ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad affrontare nella sua globalità il problema del precariato

Grazie sappiamo già che il Capo dello Stato non firmerà questo provvedimento; però, attraverso non so quale alchimia procedurale, si ritiene di approvare queste norme sapendo che esse sono radicalmente incostituzionali. Si dice: oggi le approviamo e poi con una norma le abroghiamo. Noi siamo contrari a queste procedure che si possono definire di vera alchimia regolamentare.

e assunti in servizio vengono fatte salve. Sennonché, il concorso al quale parteciparono questi candidati è stato annullato con provvedimento definitivo

così come il giudice non può sostituirsi al legislatore inventando una norma che il sistema non contiene, del pari il legislatore non può far vivere un provvedimento che è stato annullato dal Consiglio di giustizia amministrativa L'articolo 97 della nostra Costituzione stabilisce che al pubblico impiego si accede attraverso un pubblico concorso. Se il pubblico concorso è stato annullato - tanto che è in corso un giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione - non si comprende come si possa far rivivere un concorso che è stato espunto dal nostro ordinamento. Voler insistere caparbiamente su una norma palesemente incostituzionale, perché scardina il sistema armonico disegnato dai costituenti, è francamente incomprensibile.

La pretesa di voler far vivere uno strumento concorsuale travolto

all'armonia costituzionale che assegna alle decisioni della magistratura un valore vincolante anche per il legislatore, a cui si impedisce di intervenire a disciplinare quei diritti che siano stati già esaminati dalla giustizia amministrativa con provvedimento definitivo e che hanno determinato un annullamento del concorso. Nella sostanza, quindi, si è tutti d'accordo nel ritenere che praticare la strada di approvare il decreto così com'è e poi modificarlo priverebbe priverebbe il Parlamento di una sua funzione sovrana. Esiste o no un profilo di costituzionalità? Se esiste, l'Assemblea ha il dovere di apprezzarlo e decidere Non può l'Assemblea voltarsi dall'altra parte, sapendo che esiste un profilo profondo di costituzionalità, ma ignorarne e sottrarsi a una decisione coerente con quei giudizi. Sarebbe veramente contrario al rispetto che dobbiamo a noi stessi, alla funzione di legislatori, alla funzione propria del Senato e, comunque, del Parlamento non adempiere al nostro dovere di verifica della costituzionalità di un provvedimento. Quando si ritiene in maniera condivisa che il provvedimento contiene una norma incostituzionale, abbiamo il dovere di essere conseguenti, per rispetto della norma, della funzione e dell'istituzione che rappresentiamo. Per questo motivo chiedo che l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, non proceda all'esame del disegno di

Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le motivazioni che animano la questione pregiudiziale

e ne ha dedotto che egli nella sostanza condivide le preoccupazioni di costituzionalità, evocando addirittura

Il senatore Bevilacqua, con molta onestà intellettuale nei confronti della Commissione e dell'Assemblea, ha accennato e richiamato lessicalmente il comma da lei ripreso,

in ogni discussione, in ogni atto di sindacato ispettivo, tenere fuori la figura del Capo dello Stato, perché momento e garanzia di potere neutro. Il considerarlo ed evocarlo come colegislatore è improprio. So che è una scelta politica costante su molti argomenti da parte dei colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori,

alla discussione generale e alla valutazione rispetto agli altri commi, se mi permette, rovescia (appunto, da bravo avvocato) i suggerimenti e le indicazioni del relatore.

il giudice non può mai sostituirsi al legislatore e aggiunge che, di conseguenza, il legislatore non può resuscitare un concorso

*ope legis*, di assai più discreto di quello che per tantissimi anni si è consumato con cinismo sui cosiddetti precari della scuola. C'è un precedente che ha cercato di fare guerriglia nei confronti del Governo: quando il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rivendicato alla propria giurisdizione la formazione delle graduatorie provinciali degli insegnanti voleva di fatto commissariare il Governo, schiaffeggiare il ministro Gelmini, dettare i tempi ultimativi e a suo modo ricattatori, come se la giustizia amministrativa si servisse del precariato per una sua guerriglia ancora più cinica di quella che ha portato per moltissimi anni ad alimentarlo. di svolgere un'ultima considerazione. Devo dare atto al Governo, al ministro Gelmini e al ministro Sacconi di avere avuto

di presentare un provvedimento senza promettere e senza praticare, né in quest'Aula né con il sindacato, prassi di vendita delle aspettative.

rilasci di indulgenze, immissione in ruolo *ope legis*, promesse a vuoto. Questa volta si cerca di fare ordine. il decreto morisse, e morisse preventivamente, senza lasciare quegli ulteriori percorsi di ordinamento che competono al giudizio e alle valutazioni di costituzionalità (me lo consenta, senatore non sarebbe una vittoria, né per il Parlamento né per l'ordinato percorso dei giudizi di costituzionalità.

al quale forse avevano, se non qualche diritto, qualche aspettativa più che legittima. Non solo. Grazie alla sensibilità del ministro Sacconi,

Allora, senatore Li Gotti, se per la prima volta nella storia di tanti anni scolastici non si fa della gestione del negoziato più turpe, egoistico e particolaristico dei ruoli del personale l'unica questione di politica scolastica sempre all'ordine del giorno, non penso sia una vittoria delle prerogative parlamentari. Ritengo che nelle nostre prerogative parlamentari dobbiamo utilizzare l'onestà e la precisione con la quale la Commissione ci ha sottoposto il provvedimento. Poi, Poi, la maggioranza rispetterà quella «indicazione di blindatura», volta a non far morire il provvedimento. l'opposizione non farà altrettanto. Ma cedere a una cancellazione preventiva, fare irrompere fuori dalle circostanze di unità di tempo, di luogo e di azione la questione preventiva

Siamo spesso chiamati a discutere di questioni pregiudiziali in cui si ripetono stancamente alcuni elementi e si fanno affermazioni apodittiche.

prima riguarda la carenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che un decreto‑legge deve possedere ai sensi della nostra Costituzione. Credo che l'urgenza di provvedere in questa materia, al fine cioè di garantire la continuità e la qualità di un servizio essenziale come quello scolastico educativo, sia nella natura delle cose, nei fatti.

Stavo cercando di ragionare sul primo punto esposto nella questione pregiudiziale sottoposta al nostro esame questa mattina, che riguarda la carenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della nostra Carta costituzionale.

laddove parla di «consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».

dimostri, ad ogni buon conto, che l'urgenza di provvedere è davvero insita nel provvedimento, soprattutto laddove si va ad incidere su un anno scolastico in corso quale quello avviato da diversi mesi.

Il secondo punto sollevato nella questione pregiudiziale illustrata dal senatore Li Gotti riguarda la presunta violazione della legge ordinamentale n. 400 del 1988 sotto il profilo della presupposta eterogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento rispetto al suo titolo. Ebbene, credo che da una lettura attenta del provvedimento, anche alla luce delle modificazioni intervenute alla Camera dei deputati, risulti di tutta evidenza che il contenuto del provvedimento è perfettamente omogeneo e corrispondente al suo titolo: non esistono al suo interno disposizioni che riguardino altri servizi o altri settori; si tratta di disposizioni che riguardano solo ed esclusivamente, ripeto, il servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico in corso. Quand'anche vi fossero comunque dubbi e perplessità di questo tipo, come ha sostenuto egregiamente il senatore Li Gotti, il tema verrebbe poi affrontato da un'eventuale

l'incongruità dell'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies* dello stesso. Certamente la Commissione giustizia ha riflettuto a lungo su questo comma inserito nel passaggio alla Camera dei deputati e ha ritenuto doveroso segnalare un'anomalia di questa disposizione rispetto ad un sistema ordinamentale che deve garantire

proprio perché si trattava di una norma che poteva determinare l'annullamento degli effetti di provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati. Ciò non toglie però che oggi siamo chiamati proprio a ragionare su questa norma, che è una delle tante contenute all'interno di questo provvedimento, e già da un'analisi seppur superficiale del fascicolo degli emendamenti si nota come ci siano tante proposte, del relatore ma anche di altri colleghi senatori, su questo tema del famoso corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici

in qualche modo cerca di anticipare il dibattito politico in una sede non corretta. La questione pregiudiziale non può essere accolta, ma aprirà finalmente il dibattito all'interno dell'Aula su questi argomenti e anche su questa norma inserita nell'ambito del provvedimento. il dibattito politico serve proprio all'approfondimento, all'esame, all'analisi di tutte le disposizioni contenute e quindi contribuiremo tutti, ciascuno nel proprio ruolo, maggioranza ed opposizione, alla riflessione e al ragionamento su tutte le disposizioni, nessuna esclusa.

da parte nostra perché non si doveva, con il buonsenso di tutti, arrivare a questo punto della discussione con il rischio di vanificare il provvedimento. Io non sono un esperto di materie giuridiche, ma voglio ricordare, come capogruppo che ieri abbiamo dato disponibilità a votare questo provvedimento stralciando quel comma entro mezzogiorno e a riportarlo all'esame della Camera. La maggioranza ha dato all'inizio la sua disponibilità, abbiamo sospeso il dibattito

dal momento che non appare corretto un intervento legislativo diretto a determinare il mero annullamento degli effetti di provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati». Chi ha parlato prima e fa parte della Commissione giustizia si ricordi di quello che ha votato. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ho profondo rispetto e non citerò il Presidente della Repubblica, per l'autorevolezza che ha. Voglio però ricordare che stamattina il relatore ha citato questo rischio riferendosi al Presidente della Repubblica; ieri più volte l'ha citato il Sottosegretario in rappresentanza del Governo in Commissione. Io non lo citerò perché ho profondo rispetto dell'autonomia del suo ruolo, ma forse si dovrebbe rivolgere alla maggioranza. Si parla sempre di terzietà e si ricorda fin troppo giustamente che la magistratura deve applicare e non interpretare le leggi. In questo caso il Parlamento modifica un giudizio definitivo della giustizia amministrativa rispetto ad un concorso di cui autorevoli esponenti siciliani

svolto il controllo, senatrice Amati?

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

Presidente, questo è lo specchio dell'interesse che il Parlamento manifesta

La scuola è stata progressivamente deformata da una sequenza di provvedimenti occasionali, temporanei, che si rincorrevano uno dopo l'altro, che hanno svilito nel complesso il carattere della funzione docente. Non esiste scuola seria se non si riconosce alla funzione docente un carattere fondamentale nella trasmissione della cultura e soprattutto nella costruzione dialettica della capacità di esercitare il ragionamento critico. La condizione della scuola è segnata, da decenni, da una massa crescente di precari. Esiste una prima generazione di precari originari, che stiamo praticamente dimenticando e che era già numerosa, estesa, e in cui già allora ‑ parlo di un decennio fa, forse persino di più il precario tipo, o la precaria tipo, visto che c'era una maggioranza femminile, arrivava all'immissione in ruolo quasi alle soglie della pensione. Ho presenti moltissimi casi, conosciuti da me personalmente, e, poiché ho sempre vissuto nel mondo della scuola, sia pure dal lato dell'università, ne ho una cognizione precisa. Questa classe originaria di precari di prima generazione è stata soppiantata da una seconda classe di precari originatasi con le SSIS

a partecipare a corsi a pagamento, quindi onerosi, per poter fruire ad un certo punto di un punteggio. Questo punteggio, quando raggiunto, ha collocato chi usciva dalle SSIS in condizioni di prevalenza rispetto ai precari della prima generazione che, dopo aver lavorato decenni nella scuola, sono stati superati nel punteggio da quelli che uscivano dalle SSIS. Si Si è innescata in questa maniera una tipica, classica guerra tra poveri, perché nel frattempo ovviamente i docenti erano diventati o poveri o poverissimi. Questa sequenza di generazioni è stata ad un certo punto bloccata dal fatto che si è pensato di interrompere le SSIS. da 130.000 a 180.000 docenti precari (a seconda di come li calcoliamo) distribuiti in tutti i vari tipi di supplenze; essi

sono molte le scuole dove gli scolari arrivano in automobili molto più lussuose di quelle con cui arrivano i docenti (l'ho visto con i miei occhi).

perché di anno in anno i docenti vengono spediti in un posto o in un altro; vengono sostituiti, si avvicendano. Il mito originario della continuità didattica, per cui un docente poteva rimanere nella scuola per tutta la durata del corso di studi di una classe o di una sezione, è ormai un mito inesistente: la continuità didattica non esiste più, è bene saperlo. Basta fare una breve indagine sociologica per vedere che le classi di anno in anno affrontano docenti diversi:

Conosco personalmente casi di docenti che vanno a visitare gli studenti dell'anno precedente per poter godere di un minimo di calore della comunità umana.

Dove va a finire lo spessore, la dignità della funzione docente quando noi creiamo le condizioni per cui gli insegnanti sono poveri, disadattati, costretti a cambiare scuola tutti gli anni? Dove va a finire il riconoscimento dello *status* del professore? Il professore non deve essere prestigioso per come si veste o per il tipo di automobile con cui

Certo, i docenti bravi che sanno spiegare bene e costruire un rapporto con la classe abbattono qualsiasi difficoltà, ma questo è un fenomeno che dovremmo affrontare nella sua globalità.

e si vuole interrompere pure quella - hanno mantenuto con le loro lotte nei luoghi di lavoro (fabbriche e manifatture): invidia per la cassa integrazione,

Sono presenti in tribuna per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti della Facoltà di giurisprudenza della LUMSA di Roma, cui rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studi.

rappresentante del Governo, colleghi senatori, in merito al decreto-legge che intende disporre provvedimenti urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico in corso, per garantire un ombrello sociale di fatto necessario e doveroso verso i lavoratori della scuola che non hanno più la garanzia di vedersi rinnovata la nomina annuale o il contratto per le supplenze brevi, vorrei porre l'attenzione su alcuni passaggi che ritengo fondamentali oltre che positivi. Innanzitutto, a fronte di una dichiarata spesa complessiva di circa 60 milioni di euro per chiamate telefoniche e per telegrammi da parte delle scuole alla ricerca di insegnanti e personale ATA richiesti per la sostituzione di personale assente, finalmente il decreto che stiamo discutendo legittima la convocazione da parte delle scuole attraverso le caselle di posta elettronica certificata. Tale accorgimento si è reso necessario al fine di risparmiare inutili spese avvalendosi dell'utilizzo della tecnologia che certamente aiuta sia sul fronte economico che sul fronte della rapidità e tracciabilità delle comunicazioni tra l'amministrazione ed il personale della scuola. Importante risulta essere la valorizzazione del servizio prestato nello scorso anno scolastico da tutto il personale della scuola che risultava essere iscritto nelle graduatorie d'istituto. Tale decisione, oltre che valorizzare l'effettivo servizio prestato, permette un passo avanti nel riconoscimento del valore aggiunto relativo alle garanzie dell'erogazione di un servizio scolastico continuo perché premia la territorialità: la continuità didattica è un diritto degli studenti che lo Stato deve garantire, non è un *optional*. Le famiglie italiane oggi chiedono prioritariamente la stabilità degli insegnanti e questo decreto-legge viene loro incontro. Gli insegnanti non chiedono solo un ombrello sociale di tutela: chiedono soprattutto di poter mantenere una territorialità sostenibile, e questo decreto viene loro incontro. Non a caso il provvedimento ribadisce l'interpretazione autentica del comma 605 della legge finanziaria per il 2007, la stessa interpretazione che volle indicare lo stesso ex ministro Fioroni. Le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali per il biennio 2008-2010 saranno fatte secondo il principio dell'inserimento in coda, cioè sulla base dell'interpretazione voluta dall'ex Ministro, che dispose che ogni insegnante potesse scegliere una provincia in cui lavorare, e che tale scelta fosse definitiva. Sostanzialmente il Ministro chiese a tutto il personale di fare una scelta di vita. Gli insegnanti hanno il diritto di veder rispettata la loro scelta di vita professionale, che non può essere messa in secondo piano dall'introduzione di nuove regole durante la corsa. L'attuale Governo intende garantire questo diritto. Solo dopo il 2011 si potranno effettuare gli inserimenti nelle graduatorie provinciali a pettine e non prima. Voglio però a tal riguardo fare una riflessione sulla questione delle graduatorie a pettine ed in coda, questione che ha provocato ricorsi e controricorsi, decine e decine di contenziosi tra lavoratori ed amministrazione, tra lavoratori e lavoratori, tutti ad esigere, secondo il proprio punto di vista, il rispetto di sacrosanti diritti. Ebbene, mi sembra che tutti si siano dimenticati che la scuola è un servizio pubblico a favore di studenti, prevalentemente minorenni, e che essi hanno il diritto di godere della continuità educativa e didattica e di non essere danneggiati da un continuo andirivieni di docenti, anche in corso d'anno scolastico. Al centro della scuola deve stare il diritto prevalente dell'utente. Se da un lato possono essere legittime le aspettative di chi è di ruolo e si vuole inserire in graduatorie permanenti o ad esaurimento per ricollocarsi professionalmente anche su ordini di scuola diversi, dall'altro, sono inderogabili le aspettative di chi invece rischia di non vedersi rinnovato il contratto a tempo determinato; quindi la Lega Nord plaude al dispositivo che obbliga i lavoratori a tempo indeterminato ad uscire dalle graduatorie: loro hanno un lavoro sicuro, i precari no. Punto importantissimo, che la Lega Nord ha voluto in prima lettura presso la Camera, è il fatto che chi si avvale della legge n. 104 del 1992 nel momento in cui chiede l'inserimento in diverse graduatorie provinciali dovrà trasmettere alle autorità scolastiche delle province richieste, la certificazione medica originale comprovante le condizioni fisiche personali o familiari che determinano il diritto ad usufruire dei benefici concessi dalla legge n. Non solo: a decorrere dal 2009, se sussistono motivate ragioni oppure a campione, le autorità scolastiche delle province richieste dal personale scolastico potranno chiedere accertamenti sulle certificazioni relative Tali accertamenti saranno svolti presso ASL diverse da quella che ha rilasciato la certificazione stessa. A fronte delle numerose polemiche circa la regolarità di tutte le certificazioni di invalidità presentate in sede di richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali e del fatto che esse determinano posizioni posizioni in graduatoria di privilegio, come è giusto che sia secondo la legge, si rende necessario fugare dubbi e polemiche; si rende necessario che lo Stato sia garante della legalità e della correttezza di tutte le operazioni che riguardano i propri dipendenti. In buona sostanza, se c'è chi ha imbrogliato, sia smascherato e si attenga al rispetto non solo delle leggi: soprattutto, al rispetto dei colleghi di lavoro che risultano essere danneggiati nei loro diritti fondamentali. Altra novità introdotta dal decreto-legge è quella che riguarda le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale, somme che sono rimaste inutilizzate negli ultimi tre esercizi finanziari consecutivi, comprese quelle erogate fino al 31 dicembre 2009. Ecco, questi soldi dovranno essere restituiti allo Stato. La Lega Nord ritiene che sia giusto attribuire finanziamenti alle scuole a fronte dell'adesione a progetti educativi e didattici a carattere nazionale volti all'arricchimento dell'offerta formativa. È corretto che i progetti debbano essere attuati dalle scuole e i finanziamenti debbano essere utilizzati per tali progetti. Diversamente, è giusto che le scuole restituiscano i fondi inutilizzati, che attualmente formano risparmi di bilancio che in realtà non sono tali. Riteniamo importante che tali soldi debbano essere assegnati alle scuole statali per le spese di funzionamento. Positiva è l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della legge finanziaria per il 2007, finalizzata anche agli interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria, per la valorizzazione del merito degli studenti e per il potenziamento delle innovazioni tecnologiche. La Lega Nord, pertanto, ritiene che il decreto oggi in discussione sia globalmente positivo sia nei confronti delle istanze dei lavoratori precari, sia nei confronti delle istanze degli studenti e delle loro famiglie,

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, il provvedimento oggi in esame presenta una serie di problemi generali a mio avviso assai gravi. Tre sono le principali criticità del testo in esame: la parzialità dell'intervento; il problema delle pronunce della giustizia amministrativa in relazione ai ricorsi dei lavoratori avverso il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 infine, la mancanza di fondi. Per quanto concerne il primo problema, il provvedimento in esame riguarderà solo una minima parte dei lavoratori precari della scuola: il 10 per Il numero dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 ammonterebbe infatti a circa 10-12.000 unità, a fronte di una platea di lavoratori precari stimata in 250.000 unità. Nell'anno scolastico 2008-2009 risultavano occupati nelle 10.749 istituzioni scolastiche del nostro Paese 704.891 docenti e 167.123 personale ATA

A questo numero occorre aggiungere tutto il personale precario, impegnato in supplenze temporanee per la sostituzione dei colleghi assenti, quantificabile in circa 50.000 lavoratori. Il meccanismo previsto dalla cosiddetta norma salva precari inevitabilmente finirà per creare delle anomalie nelle graduatorie, in quanto rimarrà scoperta tutta un'altra area di precari che l'anno scorso non hanno avuto un incarico annuale e che risultano quindi fuori da ogni meccanismo. Connessa al problema delle graduatorie è pure la norma contenuta nel comma 4-*ter* dell'articolo 1. L'introduzione dell'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*,della legge finanziaria 2007 comporta il divieto dell'inserimento cosiddetto a pettine (cioè in base al proprio punteggio effettivo) di coloro che abbiano chiesto di essere inseriti nelle graduatorie delle tre Province oltre a quelle di appartenenza. Tale disposizione era già contenuta nel decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 ma, su ricorso dei lavoratori, la sua efficacia è stata sospesa dagli organi di giustizia amministrativa che hanno ordinato di ripristinare l'inserimento a pettine dei ricorrenti. Ora, anziché applicare quanto stabilito dalla giustizia amministrativa si tenta, attraverso il comma 4-*ter*, di aggirarlo *ex lege*. A ciò si aggiunge un provvedimento di segno contrario, ma ugualmente vergognoso, quale quello contenuto nel successivo comma 4-*quinquiesdecies*, riguardo la posizione giuridica dei candidati dei concorsi a posti di dirigente scolastico assunti in servizio. Il comma dispone, infatti, che l'annullamento di atti delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del regolamento 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano stati assunti in servizio. Una vera e propria sanatoria, ancora una volta a dispetto di quanto deciso dagli organi di controllo. Per quanto attiene ai fondi per le supplenze, non ci sono risorse aggiuntive da parte del Governo, ma viene tutto demandato alle Regioni. Le supplenze brevi sono pagate con i fondi degli istituti, ma gli istituti, per effetto dei tagli di risorse, non dispongono di fondi sufficienti. Lo Stato chiede alle Regioni di supportare questo meccanismo con risorse proprie al fine di creare nuove opportunità per i precari, come previsto dall'articolo 1, Tuttavia il provvedimento in esame, pur rispettando il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, non prevede la necessità di un coordinamento attraverso la Conferenza Stato-Regioni dei vari interventi regionali. La mancanza di un tale coordinamento è stata denunciata dalla maggioranza degli assessori regionali all'istruzione. la scelta della stipula di accordi bilaterali tra il Ministero dell'istruzione e le singole Regioni ha creato inevitabili disparità per quanto riguarda le risorse messe in campo per risolvere il problema dei precari della scuola. I primi protocolli d'intesa con il Ministero rivelano infatti differenze di trattamento tra le Regioni, le quali procedono in ordine sparso a seconda delle risorse a loro disposizione. Il Governo tradisce così il patto alla base del federalismo fiscale secondo cui, per i servizi essenziali, quali sanità, istruzione e trasporti, si impegnava a garantire parità di diritti: signor Sottosegretario, Siamo molto distanti da quello che doveva essere un provvedimento di aiuto al mondo della scuola; il Governo taglia miliardi di euro alla scuola pubblica statale, scaricando sulle Regioni e sull'INPS i costi dei licenziamenti delle precarie e dei precari della scuola. Questa maggioranza, ancora una volta, non propone forme di investimento in favore delle precarie e dei precari, non prevede alcun tipo di estensione degli ammortizzatori sociali a chi ne è escluso, e neanche ne prolunga la durata o ne incrementa l'entità, ma sembra volere, al contrario, accentuare la precarizzazione del personale docente e avviare la la regionalizzazione del sistema scolastico nazionale. È quindi davvero incredibile che si continui a parlare di provvedimento salva precari, stigmatizzato come scellerato e irresponsabile dallo stesso Coordinamento precari scuola (CPS) a livello nazionale, quando in realtà va esattamente nel senso opposto alla salvaguardia dei lavoratori della scuola.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, i nostri insegnanti stanno vivendo una realtà difficile, che proverò a spiegare. Con la trasformazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti precari in graduatorie a esaurimento, avvenuta nel 2007, le graduatorie sono state chiuse con l'intenzione di esaurirle, ossia di assumere in tempi relativamente brevi tutti gli iscritti. Contestualmente, fu posta la condizione che i docenti scegliessero definitivamente la Provincia di inclusione, senza possibilità di cambiarla, se non inserendosi in una nuova Provincia in coda. Quest'anno, in conseguenza di alcune sentenze del tribunale amministrativo, il Ministero dell'istruzione ha dovuto offrire la possibilità di scegliere altre tre Province, ponendo però il limite dell'iscrizione esclusivamente in coda. Migliaia di insegnanti, soprattutto di quella parte del Paese dove gli esuberi nel mondo della scuola (vittime delle assurde promesse di una classe politica che è poco definire irresponsabile) superano ogni fantasia, dopo aver scelto le nuove Province, hanno presentato ricorso al TAR, per ottenere l'inserimento a pettine (cioè scavalcando chi magari è da tempo in graduatoria ma con un punteggio inferiore) oltre che nella propria Provincia, anche nelle altre tre. tradotto, significa che i docenti precari, che da anni lavorano in una certa zona, si vedranno sorpassare da un numero esagerato di docenti provenienti da altre parti d'Italia. Addio così speranze di raggiungere il ruolo o, in assenza di esso, almeno il minimo di continuità didattica che si ottiene lavorando per più di un anno di seguito nella stessa scuola. Va sottolineato che a essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del Centro-Nord non sono soltanto docenti del posto, ma anche colleghi meridionali, che rischiano di vedersi sorpassare dai nuovi arrivati dopo avere per anni lavorato nelle Regioni padane, magari lontano dai propri affetti. Non si tratta quindi di una polemica Nord-Sud, ma di difesa legittima di diritti acquisiti e sudati. È in questo senso che la consideriamo una battaglia della Lega Nord. L'inserimento a pettine dei ricorrenti attuali, e di quelli che potrebbero venire dopo di loro, lede il diritto ad avere un'occupazione, esercitare la propria professionalità e raggiungere l'agognata assunzione a tempo indeterminato di chi nel 2007 ha fatto la sua scelta. Da qui il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire con legge dello Stato, che annulla le sentenze del TAR, imponendo che i supplenti siano inseriti nelle graduatorie secondo le modalità precedentemente stabilite dal Ministero. In pratica, per il periodo 2009-2010 è il blocco dei trasferimenti. Rimane però il problema del 2011, quando ci si potrà spostare in un'altra Provincia col riconoscimento del punteggio, spesso in certe zone acquisito in maniera tutt'altro che cristallina. Ecco allora la nostra decisione di presentare un ordine del giorno, che il Governo si è impegnato a trasformare a breve in un atto concreto, con cui chiediamo, nel caso di trasferimento di Provincia, la revisione dell'attribuzione dei punteggi. inoltre, a partire dalla prima integrazione delle suddette graduatorie ad esaurimento, che i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado dovranno essere valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio che, in mancanza di tale certificazione, non potrà essere valutato. Puntiamo in questo modo a stoppare il fenomeno dei docenti che figurano aver lavorato, pur non avendo in realtà mai messo piede a scuola (notoriamente ci sono docenti che pagano per avere la certificazione di servizio), e quello dei docenti che lavorano, gratis o quasi, e senza contributi, pur di avere il punteggio. Attenzione, questo è solo il primo passo, perché gli insegnanti rispettosi delle regole - che dal 2011 rischiano di trovarsi sulla strada - chiedono a gran voce la completa verifica della veridicità degli esorbitanti punteggi acquisiti da certi colleghi. Il malessere dei supplenti onesti sta incrinando anche il fronte sindacale, fino a ieri sostenitore a oltranza della scuola centralizzata. C'è già chi chiede l'istituzione di «graduatorie regionali per gli insegnanti», un albo regionale dove chi si iscrive, indipendentemente dal luogo di nascita,

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Sottosegretario, dopo un anno e mezzo di questa legislatura avrei voluto parlare nell'Aula del Senato della scuola pubblica, della scuola di cui hanno bisogno questo Paese e i ragazzi negli anni 2000, nella società della conoscenza, nel mondo globalizzato e quindi della riforma profonda della scuola. Avrei voluto parlare in particolare della riforma della scuola superiore, della formazione del personale docente, del reclutamento. Avrei voluto parlare di come si valorizza il merito degli insegnanti e degli studenti, di come si attua l'obbligo di istruzione e sono definiti i livelli essenziali di saperi, di conoscenze e di competenze che i ragazzi devono raggiungere all'interno del percorso dell'obbligo di istruzione, e così via, delle tante scelte fondamentali per il futuro della scuola, dei ragazzi e del nostro Paese. Invece, ancora una volta - ma ormai è accaduto tante volte - attraverso un decreto-legge siamo chiamati ad affrontare esclusivamente le situazioni di emergenza: far fronte, attraverso decreti e norme che si affastellano in modo del tutto disorganico, ai tagli imposti dal Governo, dal ministro Tremonti ed accettati dal ministro Gelmini. questo sia il tratto caratterizzante di tutta la conduzione del Ministero dell'istruzione da parte del ministro Gelmini e complessivamente del Governo Berlusconi: tagli, annunci, *spot* pubblicitari, ma nessun processo di riforma.

Questa finanziaria triennale ha comportato per l'anno scolastico in corso il taglio di 42.100 docenti e 15.400 ATA,

Eppure, non vi è stata una reazione sufficientemente forte e i precari nella loro lotta non sono stati adeguatamente sostenuti di fronte a questo vero e proprio dramma sociale. Il ministro Gelmini ricorda che alcuni insegnanti sono andati in pensione.

quali spesso vi sono ragazzi disabili (a volte, più di uno), stranieri, con disagi o difficoltà di apprendimento: su queste classi, a partire dalla scuola elementare, si è tagliato completamente ogni compresenza. Ricordo che nella scuola elementare l'inglese non è più insegnato da insegnanti specializzati (o

che prevede in tre anni l'assunzione di 150.000 docenti e di 30.000 ATA: si tratta di una vera e propria operazione di stabilizzazione del personale docente e non docente

Vorrei sapere dal sottosegretario Pizza qual è l'intenzione vera del Governo rispetto al mantenimento delle graduatorie, come si intende procedere sulla formazione in ingresso e soprattutto sul reclutamento del personale docente. un esempio. Nel provvedimento in esame si riconoscono i punteggi anche per quei docenti che quest'anno non avranno l'incarico di insegnamento qualora siano inseriti negli accordi fatti tra il Ministero e le Regioni. punteggio? Si intende continuare a prorogare *sine die* le graduatorie cosiddette ad esaurimento? Si intende mantenere questa modalità di reclutamento

professionale, attraverso accordi - tra l'altro privi di un accordo quadro di carattere generale - che sono stati stipulati da varie Regioni le quali integrano,

sono stati i provvedimenti dei TAR e c'è stato persino il commissariamento del Ministero della pubblica istruzione perché non dava attuazione alle numerose sentenze dei tribunali amministrativi. Devo dire che è uno straordinario pasticcio che questo Governo ha realizzato proprio perché non ha operato coerentemente con quanto la legge finanziaria prevedeva, ossia la stabilizzazione. Il ministro Fioroni aveva aperto la finestra della mobilità

Quindi, parlare di soldi non spesi suona assolutamente come una beffa nei confronti di dette scuole che stanno chiedendo alle famiglie di portare da casa persino i gessetti o la carta igienica, ossia gli strumenti fondamentali per la vita della scuola stessa, perché non hanno i soldi per pagare. dalle scuole il Sottosegretario sa bene che è per un meccanismo di relazione tra il Ministero e le scuole stesse. Da ultimo credo sia assolutamente inaccettabile che per decreto - quindi attraverso un atto di carattere legislativo - si annulli la validità di un atto definitivo della giustizia amministrativa. Ciò è tanto vero che il Governo sta trovando, con un *escamotage*, una soluzione per annullare questa norma. Quindi, chiede al Parlamento, attraverso un atto che lo svilisce completamente, di approvare ciò che non è approvabile e che il Governo stesso ha già proposto di cancellare.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, al di là degli aspetti tecnici che poi illustrerò molto sinteticamente, credo che dobbiamo svolgere un ragionamento molto più ampio: è in atto, con questo Governo, una importante riforma della scuola. Sappiamo che negli ultimi trent'anni la scuola è stata considerata una sorta di ammortizzatore sociale.

di tutti quelli dei Paesi occidentali. Si è quindi investito sulla quantità e non sulla valorizzazione professionale.

Nella scorsa finanziaria il Governo ha voluto razionalizzare gli organici della scuola italiana, prevedendo tagli certamente importanti, ma voglio aggiungere che tagli

su un sistema del tutto identico al precedente e quindi era un po' come un vestito che rimaneva lo stesso, ma il soggetto che lo indossava era cresciuto di peso

per distribuire queste risorse premiando i docenti preparati e di qualità. Questo è un passaggio assolutamente importante. È logico che per qualche anno anno i pensionamenti siano inferiori ai tagli di organico, soprattutto per quest'anno, perché poi la situazione è destinata a migliorare sensibilmente nei prossimi anni e i dati del Ministero della pubblica istruzione dicono che già nel prossimo anno dovrebbe esservi sostanzialmente una equivalenza

che serve anzitutto ad evitare un pregiudizio a coloro che avevano svolto supplenze annuali e poi, grazie ad un importante emendamento approvato alla Camera che citerò subito, anche ad altri precari, impedendo che rimangano senza una retribuzione

quegli insegnanti precari che hanno svolto un insegnamento con contratto annuale nell'anno precedente ovvero, in base all'emendamento della Camera, una supplenza di 180 giorni.

tuttavia rimanessero esclusi da queste supplenze annuali, e che dovrebbero essere peraltro in numero assai limitato, di partecipare a progetti regionali finanziati con fondi dell'Unione europea. Ovviamente, tutti quei precari che rimanessero a casa per il prossimo anno scolastico godranno - questo è scontato - del 60 per cento dell'indennità di disoccupazione.

avranno comunque riconosciuto il punteggio ai fini delle graduatorie. Credo che tutto questo denoti un comportamento responsabile, certamente doloroso per alcuni, lo dico con grande franchezza, ma il Ministero si è comportato in modo responsabile e le prospettive per l'avvenire sono quantomeno rassicuranti.

statale, cioè senza che venissero pagati i contributi, in sostanza accordandosi in modo truffaldino con una scuola che fingeva l'assunzione soltanto al fine di guadagnare punteggio. Questa è la situazione.

dei nostri docenti. Ci sono 230.000 precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ci sono 130.000 precari con contratto annuale, delle cifre veramente imponenti. Il problema del precariato è un problema vecchio, lo sappiamo perfettamente, deriva da un sistema unico in tutto l'Occidente, da un sistema inventato nella prima Repubblica, proprio da quelle magagne e da quelle carenze che avevo prima evidenziato. Ritengo però indegno di un Paese civile che famiglie che si reggono su uno stipendio che peraltro è già assai modesto non sappiano ogni anno quale sarà il proprio futuro. Ritengo che il sistema del precariato, come sistema in sé, debba essere eliminato una volta per tutte; ritengo anche che sia indegno di un Paese civile che si seguano, come hanno seguito i Governi del passato, logiche levantine per cui conviene di più pagare dieci mesi un insegnante che svolge un servizio per tutto l'anno. Il ministro Fioroni aveva a suo tempo presentato un piano di assunzioni che non solo era limitato, ma che non era coperto, era l'ennesima truffa della politica che alla vigilia delle elezioni dice: «vi assumeremo tutti e non aveva stanziato le risorse per coprire questo impegno. Vi chiedo che nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria si faccia una programmazione annuale,

Ringrazio anche il Governo di aver accolto come vincolante un mio ordine del giorno, firmato anche da altri colleghi, con cui si chiede che si avviino dei prepensionamenti per favorire il *turnover*, per consentire cioè a quegli insegnanti anziani, che magari sono anche ormai demotivati, a cui mancano due anni per poter andare in pensione, di andare in pensione anticipatamente.

Ripresenteremo questo emendamento in un prossimo provvedimento. Abbiamo l'assicurazione del Ministero dell'economia e delle finanze che questo provvedimento potrà andare in porto. Crediamo che sia un fatto di civiltà risolvere il problema del precariato. Il decreto-legge in contingente temporanea ad una grande riforma della scuola come quella che questo Governo sta iniziando ad attuare farò un intervento tematico e parzialmente diverso da quelli che sono stati svolti fino a questo momento. Visto che si parla di precarizzazione di insegnanti, di immissione in ruolo e di continuità del servizio scolastico, credo sia anche utile parlare degli insegnanti di religione. Non parlerò dell'ora di religione e di crocifisso; parlerò però di diritti e di doveri degli insegnanti di scuola pubblica e di separazione tra Stato e Chiesa.

è stata prevista l'entrata in ruolo con un concorso di 15.000 insegnanti di religione più altri 10.000. Tra i titoli richiesti c'è un riconoscimento, certo, della Curia, però c'è un appunto sicuramente più interessante, ossia che i circa 25.000 insegnanti di religione, al al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dallo Stato italiano: formati e indicati dall'autorità religiosa ma retribuiti da quella statale. C'è un'evidente discriminazione di tipo lavorativo, tant'è che è aperta una questione con la Comunità europea per quanto riguarda una direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In questo caso professare una religione diventa una discriminante in senso positivo. Esiste anche una discriminazione economica di retribuzione, sempre in positivo, per gli insegnanti dell'ora di religione. Ho presentato l'ordine del giorno G101, con il collega senatore Marco Perduca,

a quella del Concordato, ma quando si parla di diritti di lavoro, di diritti anche degli insegnanti, credo sia utile specificare come nella scuola pubblica la separazione tra lo Stato e la Chiesa debba essere evidente anche a partire dal trattamento degli insegnanti. Quindi, pari diritti per tutti gli insegnanti, a prescindere dalla materia che viene insegnata, in termini sia di retribuzione che di assunzione, senza appunto discriminazione di tipo religiosa; che professare una religione

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, sia introdotta una previa intesa in sede di Conferenza unificata per la promozione dei progetti ivi previsti, in particolare considerando che la norma affida alle Regioni il corrispondente onere finanziario. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.27, 1.34, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.55, 1.77, 1.78, 1.79, 1.83, 1.80, 1.81, 1.82, 1.86, 1.90, 1-*quinquies*.0.2, 1.35, 1.87,

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.54 e 1.56. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 1.94 e 1.92, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

contrarietà sulla restante parte. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti». i colleghi che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, gli ordini del giorno G101, G102 e

precarietà e insicurezza del posto di lavoro, ciò che caratterizza la condizione di queste persone è il fatto che questi anni non sono assolutamente validi

nella scuola italiana di questo personale, adatto anche alle nuove metodologie didattiche. Coloro che sono supplenti da anni

che i contratti a tempo determinato, stipulati con il conferimento delle supplenze, possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel caso - con una norma aggiunta alla Camera - si tratti di immissione in ruolo, con l'emendamento in titolo chiediamo anche che vi sia l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dalla legge n. 312 del 1980, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo, docente e non docente. È un'affermazione di principio molto concreta che mira a rendere pienamente operativo, e ripristinato, il diritto al lavoro che riguarda le persone con contratto a tempo determinato che vengono immesse in ruolo.

si riferisce soprattutto

dà una indicazione curiosa e ci dice che l'amministrazione scolastica può prevedere la collaborazione con le Regioni, su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni, per lavorare intorno al tema dell'adempimento dell'obbligo scolastico; un tema centralissimo della vita della scuola, tema centrale nella Costituzione.

Si indica per queste attività il profilo delle attività straordinarie - ripeto - con lavoratori precari, con risorse messe a disposizione dalle Regioni, Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo punto: siamo su un provvedimento che ha a che fare - lo si dice nel titolo - con la continuità del servizio scolastico, quindi con la stabilità del personale docente. Sappiamo che questo provvedimento non affronta adeguatamente il problema e non lo risolve. La spia di questa inadeguatezza risiede nel fatto che sull'obbligo scolastico, uno dei punti importanti, si va ad intervenire con una normativa del tutto precaria, di respiro brevissimo, del tutto insufficiente ad affrontare un problema che è il buco nero della scuola italiana: dai 13 ai 16 anni abbiamo il problema degli abbandoni. È come se si dicesse che l'obbligo costituzionale di fare in modo che l'obbligo scolastico diventi effettivo nel nostro Paese non è più in capo allo Stato ma diventa quasi residuale ed affidato in un certo senso alla buona volontà delle Regioni; contrario, ci sarebbe bisogno di un impegno prioritario del Governo per sostenere le scuole, gli enti locali e le Regioni in questa grande strategia di rafforzamento del servizio di istruzione in tutto il Paese, soprattutto nell'arco temporale della scuola dell'obbligo. In particolare vorrei segnalare che questo profilo minimalista si inserisce in un contesto in cui in questi giorni si evidenziano anche le sofferenze più acute di una scuola e di un obbligo scolastico abbandonati sostanzialmente dal Governo perché in quelle norme c'è anche l'obbligo scolastico per tutti, secondo l'articolo 3 della Costituzione, in particolare per i soggetti con disabilità. Oggi siamo di fronte ad una situazione in in cui, di fronte all'aumento di 4.000 disabili nella vita scolastica del nostro Paese, c'è il taglio di almeno 500 docenti. Quindi, come si fa a pensare che gli interventi sull'obbligo scolastico possano essere di carattere straordinario, durando dai 3 agli 8 mesi con personale precario con soldi (che forse non ci sono) del tutto insufficienti ed affidati alle Regioni. Vorrei invece dire - e concludo, signora Presidente - che ci vuole ben altra strategia, a partire innanzitutto da un rapporto organico, istituzionalizzato ed efficace con la Conferenza Stato-Regioni. Di nuovo è la Costituzione che ci richiama a questo: è il Titolo V. Bisogna che gli interventi, anche previsti in questa forma minimale, siano di un sostegno robusto della Conferenza Stato-Regioni: devono essere valorizzate ampiamente, secondo il riconoscimento dell'autonomia territoriale, le autonomie delle Province e dei Comuni; abbiamo bisogno che siano valorizzate le istituzioni scolastiche dell'autonomia intorno ai progetti didattici ed educativi, perché devono essere loro coloro che analizzano i bisogni ed indicano le risposte.

al tema drammatico dell'evasione dall'obbligo scolastico. Occorre poi una grande strategia politica, che coinvolga non solo le istituzioni ma anche i territori, le loro espressioni vitali, le organizzazioni economiche e sociali, il volontariato e l'intero Paese.

vuole dare un'indicazione positiva: obbligo scolastico, obbligo di istruzione, obbligo per i ragazzi di non perdere le opportunità, a cominciare dai primi anni di vita.

disinvestendo, come si sta facendo, non nell'abbandono ma nel sostegno, nella promozione del bene più importante di cui il nostro Paese dispone: il sistema scolastico italiano. Se non l'avessimo ancora capito, il più recente documento della Banca d'Italia ci dice il rafforzamento dell'istruzione fa aumentare il PIL. Quindi, se siamo interessati a tale risultato dobbiamo capire che occorre partire dalla leva principale, quella del sistema di istruzione del nostro Paese.

con un corrispondente taglio del personale docente e ATA di 132.000 persone. Proponiamo con tale emendamento una consistente riduzione di questi tagli: essi sono la causa del

con la relativa copertura finanziaria. È chiaro che la stabilizzazione del personale della scuola è già un obbligo legislativo che la legge finanziaria del 2007 aveva posto in carico al Governo; obbligo quantificato in 150.000 docenti in tre anni, con *tranche* di 50.000 docenti ogni anno; un obbligo che questo Governo ha completamento disatteso. Ora, l'istituzione di tale fondo può contribuire a rafforzare e rendere operativa questa scelta e permetterci di conseguire l'obiettivo fondamentale di dare più serenità e stabilità al personale docente e, conseguentemente, garantire la qualità scolastica attraverso la continuità didattica, perché tutti conosciamo benissimo il valore della continuità didattica rispetto all'apprendimento dei ragazzi ed anche rispetto alla costruzione di un'adeguata relazione educativa tra docenti e ragazzi.

1.27, che può determinare davvero quel salto di qualità nella gestione del personale della scuola e può permettere di conseguire l'obiettivo, che tutti condividiamo, di portare ad esaurimento le graduatorie e di inserire un'innovata modalità di formazione in ingresso del personale docente e di reclutamento dello stesso. Finché non si arriva al compimento di questa operazione, è evidente che tutte le affermazioni del Ministro che riguardano l'innovazione nel reclutamento del personale docente e nella sua formazione sono soltanto degli *spot* privi di contenuto operativo.

una questione di principio e di rispetto delle regole democratiche. La norma introdotta dal decreto è, infatti, una norma che annulla i procedimenti di impugnazione, che già troppo spesso hanno visto soccombere il Ministero, rispetto alla sua decisione di inserire i docenti in coda invece che attraverso la procedura, *media*, a pettine. La norma nasce come semplice interpretazione del volere del legislatore di allora, ovvero del legislatore che ha approvato la finanziaria per il 2007. A differenza dei colleghi dell'attuale l'abbiamo approvata; immagino di poter sostenere che essa non vuol significar altro nel suo dispositivo, così come peraltro già ripreso più volte dai TAR, che i docenti, durante le procedure di integrazione delle graduatorie, devono vedersi riconosciuto il punteggio raggiunto in tutte le tre province per le quali hanno prodotto

degli errori fatti dagli uffici (come nel caso in questione e in quello del concorso per dirigenti scolastici) o, come accade sulla giustizia, dai politici (come nel caso della prescrizione breve). L'Italia dei Valori si batte affinché i docenti si vedano riconosciuto il diritto al proprio punteggio e si batte con ancora più forza perché sia riconosciuto quel diritto alla giustizia che lo Stato deve riconoscere in nome del popolo italiano e che lo stesso Stato - a causa di un Parlamento che risponde ciecamente di sì alle richieste del Governo - finisce per negare a quei ricorrenti a cui aveva chiesto di proporre un ricorso in quel determinato modo. Siamo alle solite: prima si decide di giocare e quando ci si accorge che l'avversario, ovvero i cittadini, è in condizione di vincere, allora si cambiano le regole del gioco. L'Italia dei Valori starà sempre dalla parte dei cittadini.

nella sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. Sono certo che tra i vincitori ci sono anche e soprattutto docenti preparati; noi vogliamo dirlo con forza, perché non si tratta di un accanimento nei confronti dei vincitori: l'Italia dei Valori ne fa una battaglia di principio, e chiede l'annullamento del concorso e il suo riespletamento. Per questo motivo proponiamo la soppressione di questa disposizione o la sua sostituzione, e al riguardo abbiamo un altro emendamento, con questa sanatoria il problema che fa riferimento all'annullamento del concorso.

dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie che nell'anno scolastico 20082009 fosse destinatario di contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, abbia avuto una supplenza di 180 giorni e per l'anno in corso non abbia contratto analogo. Riteniamo - come ho già detto in discussione generale - che questa disposizione restringa troppo la platea dei beneficiari e per questa ragione abbiamo presentato anche altri emendamenti

Per quanto attiene infatti ai fondi per le supplenze, non ci sono risorse aggiuntive da parte del Governo, ma viene tutte demandato alle Regioni. Le supplenze brevi sono pagate con i fondi degli istituti, ma questi, per effetto dei tagli, Lo Stato chiede alle Regioni di supportare questo meccanismo con risorse proprie, potenziando l'offerta formativa e, attraverso questa, creare nuove opportunità per precari. A questo proposito, riceviamo osservazioni da tanti assessori regionali che si sono dichiarati contrari a questo provvedimento e chiediamo che l'intera questione venga discussa dalla Conferenza Stato-Regioni.

I primi protocolli d'intesa con il Ministero rivelano infatti differenze di trattamento e le autonomie hanno proceduto in ordine sparso. L'emendamento 1.43 1.43 intende specificare che nella realizzazione dei progetti si deve ricorrere ai lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 del decreto‑legge, non «prioritariamente» ma con «precedenza assoluta». Inoltre, non convincendo l'espressione di corrispondere un'indennità di partecipazione per le prestazioni nelle attività progettuali, proponiamo di modificare il testo indicando che ai lavoratori precari coinvolti nei progetti venga corrisposto un trattamento economico in base al contratto collettivo vigente nel comparto scuola, qualificando l'attività lavorativa svolta come lavoro dipendente. Questa formulazione sarebbe perfettamente coerente con quanto prescritto nel comma 4 relativamente alla valutazione di servizio e, conseguentemente, all'attribuzione di punteggio. Prego,

Il primo è l'emendamento 1.100, finalizzato

Prego, senatore Vita. che tutti seguissimo con attenzione. Effettivamente l'emendamento 1.100 vuole dare un significato più logico ad un provvedimento che, nato per evitare in un certo senso che i precari si trovino.... Senatore Butti, ho chiesto cortesemente ai colleghi di abbassare il volume della voce. Poiché io stessa faccio fatica a sentire, ho fatto alzare il volume dei microfoni. Vi invito ad abbassare il volume della voce. VITA

ai precari, lo si deve fare in modo più coerente. Dunque, non si può riservare, perché non c'è motivo che lo giustifichi, questo eventuale recupero di cui al provvedimento solo ad un segmento molto specifico e fotografato (quasi un'istantanea), come se tutti gli altri precari fossero un po' meno cittadini precari. Il precariato non va bene per nessuno. Sarebbe stato augurabile che, come come previsto nel 2007, il lavoro precario nella scuola diventasse stabile. Tuttavia, se si affronta l'argomento, vale la pena di affrontarlo in modo che anche l'annata 2007-2008 venga considerata come valore

si vuole sopprimere il comma 4-*quinquiesdecies*; un comma - e taccio - che andrebbe letto, riletto,

sanatoria del tutto al di fuori dell'immaginabile. È un atto molto grave di cui ci assumeremmo una responsabilità assolutamente impropria ed anche un po' indecente.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010», premesso che i ristretti tempi a disposizione del Senato non consentono la modifica del provvedimento e la conseguente terza lettura da parte della Camera dei deputati, pena il rischio della mancata conversione nei termini costituzionali; considerato che il decreto-legge non esaurisce il complesso tema del precariato scolastico, fornendo una risposta essenziale nell'immediato ma insufficiente a risolvere il fenomeno nel suo complesso, impegna il Governo ad affrontare tempestivamente la questione dandole definitiva soluzione con particolare riferimento ai seguenti profili: 1. estensione anche all'anno scolastico

espletato in Sicilia, rispetto al quale abbiamo la stessa opinione dei colleghi dell'opposizione; metodologicamente ci muoviamo in maniera diversa, ma pretendiamo dal Governo un impegno ad riguarda l'«estensione anche all'anno scolastico 2010-2011 delle norme di priorità assicurate dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 134». Si tratta di quelle norme di priorità che interessano il personale precario, che ha avuto incarico fino alla fine dell'anno scolastico e ha realizzato i 180 giorni nell'anno 2008-2009.

ivi richiesti; 3. revisione dell'attribuzione dei punteggi a partire dal biennio 2011-2012/2012-2013 nel caso di trasferimento di provincia del personale docente ed educativo, prevedendo in particolare che i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado siano valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio

inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l'anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e Scienze della formazione primaria; 5. soluzione della questione del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, annullato con le sentenze nn. 477 e 478 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati, eventualmente prevedendo corsi di formazione della durata non inferiore a tre mesi per i candidati che hanno prodotto ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato o diffida all'ufficio scolastico regionale per l'annullamento degli atti concorsuali; 6. reinserimento in coda nelle rispettive graduatorie generali di merito d'appartenenza, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dei vincitori e degli idonei del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e riservato per dirigenti scolastici, rinunciatari alla nomina o che, dopo l'accettazione della stessa, non hanno sottoscritto il contratto o assunto servizio; previsione che gli stessi siano nominati sui posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale d'appartenenza e a domanda, come previsto dall'articolo 24-*quinquies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, anche nell'ambito intersettoriale ed interregionale». Questo punto riguarda quei dirigenti scolastici vincitori del concorso riservato del 2004 che, dopo aver firmato il decreto di accettazione di nomina o avendo rifiutato la nomina stessa, hanno perso il diritto a restare nelle graduatorie di merito. Riteniamo che sia giusto inserirli in coda a tutte le graduatorie, ma dando loro comunque la possibilità di diventare dirigenti, risultato la «trasformazione ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie» - sono graduatorie che riguardano l'alta formazione l'alta formazione musicale - «abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni». Questi interventi non richiedono alcun impegno di spesa. giorno impegna il Governo «a valutare misure idonee per: esaurire sollecitamente le graduatorie con definitiva immissione in ruolo dei precari della scuola attraverso un piano straordinario di assunzioni; reperire risorse adeguate ad assicurare la qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo nelle scuole paritarie». Questa seconda richiesta è più blanda perché - come si capisce - è previsto un impegno di spesa che sappiamo

Senatore Valditara, accetta

settembre 2009, n. 134, come sapete, nasce da una grave emergenza: è un tentativo, per quanto limitato, di dare dare risposta ad un problema fortemente sentito dal Governo. Il decreto-legge, quando è arrivato alla Camera, non è stato blindato; infatti profonde modificazioni, dovute proprio alla volontà del Governo di confrontarsi con l'opposizione, con tutte le opposizioni. Le modifiche che sono state sono state decise alla Camera dei deputati sono estremamente significative, soprattutto per quanto riguarda il reinserimento di una graduatoria unica e la fine dell'inserimento in coda

i testi sono migliorabili: ho sempre sostenuto che c'è la possibilità di lavorare insieme, soprattutto in un intervento come questo, che, anche se non è esaustivo, affronta il problema di migliaia e migliaia di precari, ma soprattutto si preoccupa di non perdere risorse che quanto prima saranno utili al sistema scolastico. Se non ho accettato ieri la proposta

Il Governo ritiene che non ci siano motivi di incostituzionalità, ma che si sarebbe perpetrata un'ingiustizia grave; il comma 4-*quinquiesdecies* è il frutto della modifica affrettata di un emendamento, ma soprattutto voglio ribadire che il Governo intende

per l'abrogazione del comma, così come propone nell'emendamento il senatore Giambrone.

che avrebbe portato all'esaurimento delle graduatorie: quel piano è stato mandato all'aria. Vorrei richiamare semplicemente il il dramma umano, e qualche volta anche la disperazione, di chi, dopo aver insegnato un decennio, e a volte anche più nelle scuole, e quindi aver elaborato un progetto professionale e di vita, ora si trova quella strada completamente sbarrata. Sappiamo, signora Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, che questo provvedimento è figlio di quella voragine che è stata aperta dal decreto-legge n. 112 dello scorso anno, che qui è stato richiamato e che ha prodotto tagli per 8 miliardi e mezzo di euro nelle scuole. Sono tagli insostenibili! E sapevamo anche che questo sarebbe stato l'esito, cioè un licenziamento di massa nella scuola. Vorrei richiamare l'attenzione anche su un altro fatto, ossia che nella stragrande maggioranza gli insegnanti licenziati sono donne: donne espulse dalla scuola senza tutele. Questa è la realtà che stiamo provocando. Non può dire il ministro Gelmini che con questi licenziamenti si migliora la scuola e si introduce il merito: questo per me è davvero risibile. Parliamo di insegnanti che hanno già superato la fase del reclutamento in qualche forma (che siano le SSIS, il concorso o altro) e che, avendo insegnato per anni, hanno maturato esperienza e competenza; sanno che il merito si raggiunge attraverso obiettivi, come per esempio portare gli studenti al successo formativo. Non sono cooptati senza merito, anzi credo che un Ministro dovrebbe riconoscere il ruolo prezioso svolto finora da questi insegnanti nella e per la scuola del nostro Paese. Occorre più rigore nella scuola? Certamente, ma con la formazione, creando condizioni di maggiore coinvolgimento e di serenità, una scuola più moderna,

Questo occorre fare se vogliamo davvero migliorare la nostra scuola e non portarla alla dissoluzione. Certo, non possiamo accettare la brutalità del dire «facciamo un bel taglio ed è tutto risolto», perché questo per noi è offensivo e inaccettabile. Com'è inaccettabile l'intento l'intento punitivo che percorre questo provvedimento. Penso, tra le altre cose, a quell'appesantimento burocratico che riguarda, ad esempio, l'applicazione della legge n. Di nuovo - vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi - vengono colpite le donne, tra le altre cose; a queste donne si chiede sia l'assistenza e la cura dei familiari che ne hanno bisogno,

se si immagina che i provvedimenti di emergenza debbano avere un segmento di utilizzatori preso a caso, si crea una precondizione anche per situazioni omologhe in altri provvedimenti. Il mio è un tentativo

visto il destino che ha avuto l'emendamento 1.35 che invece affrontava la materia in modo globale. Mi riferisco al famoso comma 3, ampiamente ricordato, in cui si introduce una novità abbastanza inqualificabile dal punto di vista istituzionale e del nostro ordinamento. Praticamente l'amministrazione dello Stato,

Se le Regioni non vogliono vedere sul loro territorio gli effetti socialmente insostenibili di questi tagli, possono mettere a disposizione delle risorse per attività che possono anche essere rivolte alla garanzia dell'adeguamento dell'obbligo scolastico. Con questo modesto emendamento Con questo modesto emendamento cerchiamo almeno di ridare un minimo di dignità istituzionale alla questione e di riferirci ad un accordo quadro Stato-Regioni.

se il Governo taglia e le Regioni devono mettere le risorse per coprire gli obblighi previdenziali spettanti allo Stato? È un federalismo fiscale al contrario:

Signora Presidente, non voglio aggiungere altro a quanto già detto dalla collega su questo emendamento. Mi permetto di fare una semplicissima riflessione: è stato già sottolineato che ci troviamo a dover affrontare una riforma della scuola che non parte da un progetto culturale, ma da un'esigenza di bilancio. 112 del 2008 ha tagliato le risorse, ha tagliato gli organici e prevede una *road map* - diciamo così - sulla contrazione del personale che determina la necessità di adeguare alla manovra economica di un anno e mezzo fa il sistema degli organici e del reclutamento. su sollecitazione della magistratura amministrativa e di giudicati, poco importa se cautelari o di merito, che si sono formati intorno a decisioni discutibili che il Ministero ha assunto in ordine alla redazione delle graduatorie per i cosiddetti precari.

tutti i sistemi e tutti i criteri oggettivi seguiti dal 1999 ad oggi per definire delle graduatorie basate su regole oggettive che valgano in quanto tali per tutti e costituiscano un sistema di selezione su tutto il territorio nazionale, è un altro paio di maniche. Ad esempio, l'idea

la valutazione deve essere valida per tutto il territorio nazionale, altrimenti si alimenta il legittimo sospetto che si preveda l'inserimento in coda in alcune graduatorie solo perché questo consente al Nord di selezionare in modo speciale il personale docente. Ci troviamo in questo momento a dover intervenire con un decreto-legge rispetto a una decisione che il Consiglio di Stato ha assunto qualche mese fa, quando ancora il Ministero poteva intervenire senza bisogno di emanare un decreto-legge, correggendo i decreti ministeriali legittimi che aveva emesso. Oggi interviene anche una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che in qualche mondo rende ancora più caotico il sistema, i precari una spregevole guerra tra poveri, che vedo oggi cercare il parlamentare X anziché il parlamentare Y per essere inseriti in posizione di maggiore o minore vantaggio all'interno di una graduatoria che, comunque, è destinata ad essere a esaurimento. Di questo purtroppo stiamo parlando, e le vittime, oltre agli insegnanti e ai precari, sono le famiglie italiane che si trovano nell'incertezza in merito al tipo di assistenza e di servizio scolastico che la scuola pubblica deve offrire. è, se ormai non ci meravigliamo più della circostanza che gli insegnanti pubblici possano essere considerati a tutti gli effetti dei cassaintegrati, ancorché per otto mesi; se non ci meravigliamo più neanche della circostanza che per poter prestare assistenza almeno ad una parte di questi insegnanti precari (che vengono definiti non utili nel momento in cui si deve procedere al taglio delle risorse alla scuola e a quello delle graduatorie) gli si

volevo fare una brevissima dichiarazione di voto richiamando un fatto. Quando nel 1977 è stata approvata la legge n.

Quella legge prevedeva l'abolizione delle classi differenziali e speciali. I bambini e i ragazzi portatori di handicap - oggi li chiamiamo diversamente abili, allora si chiamavano portatori di handicap

o l'assessore. In particolare, mi rivolgo solo ad una persona. Ho fatto l'assessore alla Provincia di Milano mentre faceva l'assessore al Comune di Milano Ombretta Colli. Mi rivolgo a lei perché la conosco personalmente e so che, come me, lei non vuole assolutamente tornare alle scuole speciali o alle scuole differenziali. Noi consideriamo superato quel momento; quindi, se si dimezzano gli insegnanti di sostegno e si riducono le risorse, è chiaro che quei bambini del Comune di Milano, di Bernareggio, di Catania o di Catanzaro che hanno una disabilità

quando i bambini diversamente abili avevano meno diritti all'interno della nostra società.

e vorrei ricordare un piccolo particolare. È assolutamente vero che gli educatori di sostegno sono un problema per le nostre scuole e noi, che facciamo gli amministratori locali, purtroppo lo sappiamo molto bene. vorrei ricordare che - come ha detto la collega - sono passati 32 anni dal momento in cui le funzioni vennero attribuite ai Comuni:

in determinati progetti possono usufruire anche di un ulteriore beneficio consistente in un'indennità a carico delle finanze regionali. Sarebbe giusto ampliare a tutti

che non sparisce alcun posto di ruolo, ma si permette ad una persona, che è in ruolo e magari ha una professionalità ed una competenza maggiori in un'altra classe di concorso (che ha superato), di andare in ruolo in quella disciplina, liberando un posto a tempo indeterminato nell'altra disciplina. Mi sembra che in tal modo si premi una maggiore competenza e professionalità.

Presidente, abbiamo ascoltato le parole del Sottosegretario, ma non possiamo ritirare l'emendamento

per la soluzione della questione del concorso per dirigenti scolastici - sapete già tutto perché avete respinto la nostra questione per l'annullamento degli atti concorsuali. La maggioranza e il Governo ci dicono cioè che hanno votato contro la pregiudiziale ma sono d'accordo;

che sono stati poi tradotti in fatti concreti. Di fatto assistiamo ad un provvedimento definitivo della giustizia amministrativa che viene annullato, ad una nota estremamente dura dello stesso giudizio amministrativo che chiede di ottemperare. Chiediamo giustamente ai magistrati di non interpretare le leggi

Mi sembra che la credibilità davanti al Paese che ci sta ascoltando sia nulla. Ripeto l'appello che abbiamo fatto ieri:

una illegittimità ed una disparità di trattamento tra idonei e vincitori, ossia tra coloro i quali erano idonei e vincitori inseriti in graduatoria senza che avessero avuto l'assegnazione del posto ma avevano scontato positivamente un giudizio di merito favorevole rispetto ai criteri stabiliti. Questo la dice lunga sulla circostanza, proprio perché si è delegato al giudice amministrativo il compito di stabilire regole chiare e certe che valgano per tutti, indipendentemente dal colore politico del Governo del tempo e dai sindacati che riescono a fare pressione per avere determinati criteri anziché altri nella determinazione dei decreti ministeriali sulle graduatorie delle supplenze, i quali poi hanno alimentato l'indegno serbatoio del precariato. A prescindere da tutto questo, già quelle norme erano di per se incostituzionali. Non c'è bisogno ‑ collega Giambrone, lo dico con tutto il rispetto che ho per lei e per la bontà della sua iniziativa ‑ di dire una cosa ovvia, non è possibile che si intervenga con legge per sanare vizi che sono già stati consolidati in decisioni della magistratura. Ma siccome queste sono regole che dobbiamo il tempo a mia disposizione. Cerco di usarlo con parsimonia, e solo su alcuni aspetti che credo siano utili ed importanti.

per una norma che sana - ripeto - le illegittimità che sono state consumate nella redazione delle graduatorie, né per una norma che dà certezza e stabilità all'anno scolastico. Infatti prima si è creato il presupposto per l'annullamento giudiziale

Siamo d'accordo sul fatto che si debba fare qualcosa per i precari, ma certamente non ci si può mettere nelle condizioni di decidere su questi fatti a babbo morto. Questo è il senso della nostra astensione.

*relatore*. Signora Presidente, qualcuno ha fatto riferimento all'«indegna soppressione del precariato»: il precariato non lo ha costituito il Governo Prodi, né questo Ministro. È vero che il Governo Prodi aveva previsto un

il concorso, sul merito siamo tutti d'accordo e diciamo tutti la stessa cosa: il problema è che non si può pensare che questo provvedimento vada alla Camera e venga approvato Ci fidiamo di quello che promette il Governo, l'abbiamo chiesto in maniera forte e siamo convinti che il Governo darà seguito all'impegno. Ribadisco che se questo non dovesse succedere ne prenderemo atto per il futuro. Certo, e mi rivolgo al senatore Rusconi,

che ha istituito una nuova categoria: dopo gli emendamenti decaduti, quella del suicidio dell'emendamento. Vorrei rispondere con un dato semplice, ovvero che questi presidi - così parlo un linguaggio chiaro a tutti - sono in ruolo da due anni e sono pagati come presidi, mentre, se decadessero, verrebbe incaricato un dirigente a scavalco o un insegnante, che

da parte dell'azienda Marini di San Paolo, una società che alleva animali a scopo di sperimentazione, di 278 animali (la maggior parte dei quali cani di razza *beagle)*, a causa di una crisi finanziaria. Attraverso quest'asta la ditta in questione avrebbe ceduto l'intero *stock* ad altra società con la stessa ragione sociale, che avrebbe presumibilmente immesso gli animali nel mercato della sperimentazione.

si possono giudicare dal modo in cui si trattano gli animali». In queste ore, in questi giorni, nelle trasmissioni televisive considerate *top* da vari punti di vista, da «Annozero» a «Che tempo che fa» e «Porta a Porta», è venuta una riflessione, peraltro sollecitata da un intervento dell'onorevole Di Pietro abbastanza discutibile, di messa in ridicolo dell'attenzione agli animali d'affezione, quelli che molti preferiscono chiamare esseri senzienti. Dire che si fa male ad intervenire e magari a far passare la famosa Convenzione europea sul benessere animale, credo sia cosa grave e sia cavalcare l'antipolitica. Quindi chiedo un'attenzione dell'Aula e anche del Governo al fine di verificare che la vicenda che raccontavo relativa ai *beagle* sia veramente stata fermata e anche a far sì che non passi l'antipolitica sulla pelle non solo degli animali d'affezione, ma anche di quelle tante

Non vorrei che alcune reazioni zelanti (come già è accaduto relativamente ai prezzi della *buvette*) poi facciano girare in una beneficenza, che noi non abbiamo ancora potuto conoscere a chi vada, il risparmio relativamente all'abbassamento delle temperature (cosa peraltro auspicabilissima, visto e considerato che in effetti in Commissione si muore dal caldo), ma credo che vada fatto notare al «Corriere della Sera», e anche magari a qualche sostenitore dell'ENI, che proprio da quel pulpito una predica relativamente all'attenzione ai diritti dell'ambiente e al risparmio energetico non può venire per due squisite ragioni: in primo luogo, perché grazie all'insistenza dell'ENI noi siamo i partner strategici principali, riconosciuti da maggioranza ed opposizione, di almeno due dittature, una democratica, la Federazione Russa, l'altra meno democratica, la Libia; luogo, stiamo facendo prendere posizioni politiche all'interno dell'Unione europea da parte del nostro Governo contro il cosiddetto gasdotto Nabucco, dove invece i nostri partner stanno investendo per cercare di garantire all'Italia forniture di gas a prezzi di mercato e non - come dice giustamente invece il «Corriere della Sera» - a prezzi al di sopra del prezzo di mercato, perché ci approvvigioniamo dai partner strategici di cui sopra.

bensì raffreddati. Questo è un aspetto da approfondire. Pertanto, per abbassare ulteriormente la temperatura all'interno di questi ambienti occorrerebbe consumare una quantità maggiore di energia, che sembra essere proprio ciò che lei e tutti

Questo lo posso testimoniare personalmente, perché quando sono seduta al banco della Presidenza a volte fa molto freddo, oltre al fatto che c'è un vento incredibile.

Mesi fa abbiamo denunciato, a fronte del piano industriale della FIAT, l'ipotesi della chiusura dello stabilimento di Termini Imerese. Sono passati mesi

L'opera faraonica doveva essere già pronta entro il 2010, ma ancora non ne è stato realizzato neanche un metro. Inoltre, si vorrebbe sapere per quale motivo, a fronte di ripetuti richiami alla Corte dei conti, al collegio dei revisori dei conti del Comune e delle deliberazioni dello stesso consiglio comunale, volte al contenimento della spesa delle aziende partecipate, il sindaco e l'AMAT non abbiano ritenuto di adottare provvedimenti volti a consentire alle partecipate di incamerare direttamente le somme eventualmente destinate ai singoli dirigenti, alleviando così lo stato di sofferenza finanziaria nel quale versano le società partecipate.

Presidente, ritorno sul piano industriale FIAT e sulla sbagliata e ingiusta idea della FIAT di rinunciare alla sua presenza nello stabilimento di Termini Imerese. Presidente, la

nei propri Paesi. Ecco perché la questione è di grande rilevanza e merita la presenza del ministro Scajola qui in Aula, di fronte al Parlamento, per spiegare al Parlamento italiano quali sono le idee della FIAT. Sia chiaro, nessuno è contrario allo sviluppo della FIAT nel mondo, anzi. Questa è una grande opportunità e una grande risorsa, ma siamo fermamente convinti che la crescita della FIAT si può conciliare con un potenziamento della sua produzione innovativa in Italia ed anche con la sua presenza innovativa in Sicilia, nello stabilimento di Termini Imerese. Vista la rilevanza e la portata che presto si avrà nella presentazione del piano industriale, prima di annunciarlo al Paese, prima che la frittata sia fatta, il venga nel cuore della democrazia a confrontarsi con il Paese, attraverso i parlamentari. Vogliamo sapere, Presidente, quali sono le idee del Governo, quali sono i suoi indirizzi. Sia chiaro Sia chiaro che alla richiesta che ci viene fatta dal sindaco di Termini Imerese e dal Presidente della Regione di non votare gli ecoincentivi, senza un chiarimento di questo tipo, da parte dei parlamentari siciliani e da parte mia ci sarà un impegno severo e rigoroso, perché non possiamo accettare passivamente una decisione sbagliata e ingiusta, del tutto estranea a quello che i Governi di tutto il mondo stanno facendo per mantenere in piedi la produzione delle automobili negli stabilimenti nazionali. **Mozioni